Signor Presidente, con riferimento al viadotto situato al chilometro 21,665 della strada statale 691 Fondo Valle Sele, nel territorio comunale di Caposele, la società Anas ha rappresentato quanto segue. In seguito alla frana cui fa riferimento l'onorevole interrogante, il personale tecnico di Anas ha tempestivamente effettuato una ispezione sul viadotto in questione lo scorso 22 gennaio, in particolare sulla campata di scavalco alla ex strada

Sono stati pertanto registrati degli smottamenti localizzati che hanno coinvolto soltanto i terreni vegetali superficiali e che non hanno interessato alcun elemento di fondazione del viadotto né causato cedimenti sulle strutture. Anche sull'impalcato i tecnici di Anas hanno riscontrato l'allineamento dei giunti di dilatazione, cioè gli elementi di raccordo tra gli impalcati, e non hanno rilevato alcuna lesione sul piano viabile associabile a fenomeni di rotazioni o di cedimenti locali delle fondazioni. L'ispezione di Anas si è conclusa quindi senza la necessità di istituire alcuna limitazione al transito sul viadotto, poiché la struttura non è risultata compromessa dai fenomeni di smottamento verificatisi.

di Anas, si può dedurre che non ci siano stati danni strutturali al viadotto e che quindi questa sia la ragione della mancata chiusura.

utile per cercare di fare il punto su alcune questioni che penso valgano in senso generale, non specifico per il caso del viadotto in questione a Caposele. Il problema che le voglio rappresentare è il seguente. Abbiamo moltissime infrastrutture situate in contesti territoriali dove la proprietà privata è molto parcellizzata, quindi i fronti sovrastanti i viadotti e i tratti stradali

facciamo assumere alle società che gestiscono ferrovie e strade un po' di responsabilità sul tema dei fronti che stanno sopra queste infrastrutture; o il rischio è che, ogni volta, il danno non solo costi molto di più, ma sia anche particolarmente serio e grave per i cittadini. cittadini. È un caso abbastanza riscontrabile anche in questo esempio. Questa è una delle prime questioni: qual è la strategia del Governo per intervenire e garantire sicurezza, che siamo soggetti a una quantità enorme di eventi franosi? La seconda questione è la seguente. Ormai è del tutto evidente e del tutto appurato

Il punto, anche in questo caso, è capire quanto siamo stati in grado di espandere questi sistemi di sensori. Da quello che so, infatti, purtroppo questi sono ancora casi molto isolati. Faccio un esempio. Nella ricostruzione del ponte Morandi e del viadotto San Giorgio c'è stata questa precauzione, ma è chiaro che stiamo parlando di infrastrutture molto datate, che non hanno questi sistemi di rilevazione.

Sottosegretario, naturalmente la ringrazio per avermi illustrato il caso specifico e per aver tranquillizzato i cittadini, ma una visione su questo punto non la vedo ancora.

Mi auguro, però, siccome stiamo parlando di un tema serio, non solo che queste idee arrivino, ma che ci sia anche la capacità di ascoltare l'opposizione, perché su questo tema abbiamo lavorato tanto e abbiamo anche una certa esperienza e conoscenza del tema della rete infrastrutturale. Se lo vorrete,

Signor Presidente, onorevoli senatori, il senatore Parrini e la senatrice Zambito pongono l'attenzione sullo spaccio di stupefacenti effettuato all'interno della riserva naturalistica delle Cerbaie, chiedendo al Ministro dell'interno quali azioni intenda assumere per contrastare il fenomeno e supportare le iniziative degli enti locali in materia di sicurezza e lotta alla criminalità. Premetto al riguardo che l'area in questione - che si estende per circa 12.000 ettari, al confine tra le Province di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia - è oggetto di costante attenzione da parte delle prefetture competenti, che nella zona si sono verificati episodi di criminalità diffusa, in particolare reati di natura predatoria e spaccio di stupefacenti, agevolati dalla natura boschiva della zona. In particolare, la tematica nel corso del tempo è stata esaminata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Firenze ed è stata altresì oggetto di specifiche riunioni nell'ambito del Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da ultimo convocato il 17 novembre del 2022. Nel corso di tale riunione, presieduta dal prefetto di Firenze, cui hanno partecipato i rappresentanti delle prefetture e delle altre Province interessate i componenti dei Comitati provinciali e i rappresentanti delle relative amministrazioni provinciali e comunali, è stata svolta una disamina complessiva delle criticità che interessano alcune zone della vasta distesa boschiva. Alla luce delle richieste avanzate dall'amministrazione locale, sono state verificate le iniziative assunte finora e sono state approfondite eventuali ulteriori misure da intraprendere in condivisione con i rappresentanti delle comunità locali. Durante la riunione, è stata rilevata la necessità di approntare misure strutturate e sistematiche che tengano conto anche della complessità determinata dalla peculiare configurazione boschiva dell'area. emersa quindi l'esigenza di uno sforzo congiunto da parte di tutti gli attori presenti, nell'ottica di favorire un maggior coordinamento nell'attività di contrasto dei fenomeni di illegalità segnalati. Conseguentemente, nell'area in questione sono stati ulteriormente potenziati specifici servizi di controllo, con l'impiego di unità cinofile antidroga del reparto prevenzione crimine e del reparto volo della Polizia di Stato. Inoltre, all'esito del predetto Comitato interprovinciale, è stata affidata al locale Comando provinciale dei carabinieri - in virtù della capillare presenza sul territorio dei presidi dell'Arma l'esecuzione di uno specifico piano di interventi coordinati con gli altri Comandi provinciali e che prevedono il coinvolgimento delle polizie locali e della Polizia provinciale. Proprio in esecuzione del predetto piano, nel periodo tra il 17 novembre 2022 e il 22 febbraio 2023, sono stati condotti nell'area delle Cerbaie diversi servizi straordinari di controllo, con i seguenti risultati: 1.046 persone, 671 veicoli controllati, 3 persone arrestate e 13 denunciate. Nelle giornate del 19 dicembre e del 22 febbraio scorsi, sono stati organizzati anche servizi ad alto impatto grazie al supporto del 6° Battaglione Carabinieri Toscana e del Nucleo Carabinieri cinofili di Firenze. Come accennavo, già da tempo i servizi di controllo sono stati attivati nell'area in questione, tant'è che nel quinquennio 2018-2022 sono state concluse 90 operazioni antidroga, che hanno portato al sequestro di più di 700 chilogrammi di sostanze stupefacenti e psicotrope e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 119 persone, delle quali 87 in stato di arresto. I risultati conseguiti grazie a tale attività - che proseguiranno anche nell'anno in corso - hanno contribuito a restituire alla cittadinanza una maggiore percezione della sicurezza. Per quanto attiene ai presidi delle Forze di polizia nell'area in questione - con particolare riferimento ai comuni di Fucecchio, Altopascio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese - l'Arma dei carabinieri è presente con una forza effettiva di 59 unità e la Guardia di finanza con 166 unità. Per quanto concerne, infine, il ricorso al personale dell'Esercito, nell'ambito dell'operazione Strade sicure - cui si fa riferimento nell'interrogazione - evidenzio che, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, i militari posti a disposizione dei prefetti, nell'ambito del dispositivo di sicurezza in ambito provinciale, concorrono esclusivamente alla vigilanza ai siti e agli obiettivi sensibili. In ogni modo, l'attenzione resta alta. Infatti, allo scopo di favorire un maggior coordinamento nell'attività di contrasto dei fenomeni criminosi segnalati dagli interroganti e analizzare gli esiti dei servizi di controllo del territorio svolti lo scorso novembre, è stata programmata - il prossimo 15 marzo - una ulteriore riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Albano per la dettagliata risposta che ha dato. Non posso dirmi del tutto soddisfatto, anche se apprezzo l'impegno che è stato descritto e circostanziato. Infatti, la percezione che c'è sul territorio dei Comuni interessati - che riguarda quattro Province - è che si debba fare di più per passare dalle parole, dagli impegni e dall'enunciazione di propositi a fatti concreti. L'attenzione sarà anche alta, ma per ora la sensazione del territorio è di non essere stato adeguatamente fornito di un'assistenza e di una

questo compito di repressione dei fenomeni criminosi. È necessario un aiuto più continuativo, più strutturale e incisivo delle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza). Sarebbe estremamente necessario un forte e costante coordinamento tra le prefetture delle quattro Province interessate e bisognerebbe agire in maniera molto meno episodica per ottenere risultati strutturali. Fra l'altro, ci si può avvantaggiare in questo caso di una grande sensibilità delle popolazioni locali e anche dell'associazionismo locale, perché

molto importanti nel contrasto a questi fenomeni, tenendo alta l'attenzione sociale. Infine, richiamo l'attenzione della Sottosegretaria in maniera molto forte sulla necessità di supportare, con iniziative concrete e soprattutto con l'erogazione di contributi, un intervento strutturale, che aiuterebbe molto a rafforzare il presidio di sicurezza in quel territorio, e cioè il completamento della ristrutturazione dell'edificio per la tenenza dei Carabinieri di Il Comune di Fucecchio, come tutti i Comuni, è stato un'amministrazione il cui bilancio si è trovato posto a dura prova dall'emergenza Covid e da altre necessità che si sono presentate. Può fare la sua parte, ma ha bisogno che lo Stato sia Anche da questo punto di vista, chiederei maggiore attenzione e un occhio di riguardo, perché questo passo, se si compie, può davvero andare nell'interesse generale.

con riferimento all'interrogazione parlamentare in questione, sulla base degli elementi acquisiti dall'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza per tramite della Regione Campania, comunico quanto segue. Il presidio ospedaliero Sant'Anna e Maria santissima della Neve di Borgotrecase, in provincia di Napoli, afferente all'Azienda sanitaria locale 3 Sud, con delibera del direttore generale n. 221 del 17 marzo 2020, è stato dedicato all'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19. La direzione strategica, insediatasi ad agosto 2022, ha ritenuto, nella fase di discesa della curva epidemiologica

a grezzo, oggetto di lavori e di finanziamenti *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nonché di lavori già in corso di esecuzione e finanziati (lavori di completamento dell'area finalizzati alla realizzazione di 20 posti letto di terapia subintensiva), e la messa a norma dei locali del DEA attraverso un intervento a *step,* che consentirà, verosimilmente nell'arco di tre o quattro mesi, di avere a disposizione dal punto di vista strutturale-impiantistico un pronto soccorso in grado di garantire il doppio percorso Covid-non Covid, giusta deliberazione aziendale n. 1021 del 15 novembre 2022, come programmata dirigenziale (UOD) Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare. Ai fini del ripristino delle funzioni originali della struttura, sono state contestualmente avviate numerose procedure di reclutamento di personale medico sia per i reparti d'elezione, sia per l'emergenza-urgenza. Va anche detto che l'attuale numero di ricoveri e di accessi nelle strutture aziendali di pazienti con Covid ha imposto cautelativamente non solo il mantenimento dei posti letto Covid (32), ma anche la riattivazione in data 2 gennaio 2023 di ulteriori 10 posti letto letto dedicati all'assistenza dei pazienti Covid positivi. Attualmente, l'assistenza per i pazienti non Covid è assicurata dalle seguenti branche: cardiologia (10 posti letto), pneumologia (10 posti letto), medicina (10 posti letto), anestesia e rianimazione (3 posti letto). Riportati gli elementi acquisiti dalla Regione, passo adesso a svolgere le valutazioni di competenza del nostro Ministero. Il presidio ospedaliero in questione, nel rispetto dei profili di competenza delle Regioni, era stato individuato quale presidio Covid e pertanto destinato all'assistenza dei pazienti Covid attraverso l'attivazione e lo sviluppo di linee di attività quali la pneumologia e la terapia semintensiva e il potenziamento di servizi quali la medicina interna. Pertanto, appena sarà possibile, lo stesso presidio ospedaliero quale DEA di primo livello sarà ripristinato con la funzione originaria all'interno della rete ospedaliera così come definito dalla Regione Campania e contestualmente saranno garantite le discipline previste negli atti di programmazione e specifiche di una DEA di primo livello. Su tale ultimo aspetto, l'ASL ha comunicato di aver riattivato l'*iter* per il ripristino delle funzioni originarie verosimilmente in un arco temporale di quattro mesi, necessario per assicurare dal punto di vista strutturale e impiantistico un presidio che garantisca i necessari percorsi Covid e non Covid. Il Ministero della salute, fin d'ora, assicurerà il monitoraggio delle azioni dichiarate dall'ASL.

Signor Sottosegretario, lei ha detto che nel 2022 è terminato il periodo del presidio Covid e sono iniziate le pratiche anche burocratiche per cominciare a raccogliere tutte le energie e tutti gli sforzi anche finanziari per poter ripristinare il servizio di pronto soccorso. È passato un anno da quel periodo e adesso mi sento dire che appena sarà possibile,

Sono andato anche a fare visita al cantiere, insieme con il direttore generale, che mi ha accolto dopo ripetute richieste. La informo anche che la prima e la seconda volta non mi è stato possibile visitare il cantiere; solo dopo mia insistenza, ho potuto visitarlo. Ora, mi domando se non sia venuto il momento di mettere in discussione alcuni punti di tutto l'impianto del sistema sanitario nazionale, visto che un pronto soccorso un pronto soccorso DEA di primo livello - come lei ha affermato essere - in realtà non funziona come tale. Io e lei sappiamo benissimo cos'è un DEA di primo livello: non è un ospedale Covid, ma un ospedale per l'emergenza-urgenza,

un impegno reale a potenziare l'emergenza-urgenza, perché l'ospedale di Boscotrecase è solo uno dei tanti ospedali che hanno questa crisi

dedicato ai pronto soccorso; un unico procedimento strutturale non c'è stato, niente. Lei scuote la testa, onorevole Sottosegretario. Beh, stando sui territori le posso assicurare che non è cambiato niente: i pronto soccorso sono ancora oggi pieni di

anche la volontà da parte sua di monitorare, come Sottosegretario, l'andamento di questi lavori; questa è la parte che auspico possa essere poi presa veramente in considerazione. La invito a venire in quest'ospedale, che è in costruzione da quindici quindici anni. Quando parla di superfici grezze, è ovvio che le hanno dato un *report*: venga a vedere cos'è questo DEA di primo livello, altrimenti rimaniamo solamente nell'ambito delle descrizioni che le vengono date. Colga l'occasione per venire sul territorio, a Boscotrecase. Facciamo un'ispezione vera e reale, non qui in quest'Aula. Venga veramente e porti le sue parole, le parole dello Stato, a questo territorio, nell'ASL Napoli 3 Sud, che è una delle più popolose d'Italia, con un milione di cittadini residenti e 300.000 abitanti. Lo ripeto, perché non sarebbe possibile realizzare un DEA, se non ci fosse la stima degli abitanti che afferiscono a questo distretto: 300.000 abitanti da oltre un anno non vedono la possibilità di avere il ripristino del pronto soccorso. Offro

Signor Presidente, garbatamente, nel merito della questione delineata, mi collego dicendo che forse avrò sbagliato io nel comunicare al collega Mazzella che che riporto ciò che mi viene detto dalla Regione Campania. Lei sa meglio di me e mi insegna che la riforma del Titolo V della Costituzione porta il governo e la *governance* regionale in capo alle Regioni.

nel suo intervento, perché la conosco e so che è una persona assolutamente propositiva, e sarò con lei a verificare lo stato di attuazione, ma anche di salute della rete ospedaliera campana, partendo dal presupposto che già lo faccio di mio: giro per gli ospedali del Nord, del Centro e del Sud e non avrò difficoltà

ha comunicato al Ministero le informazioni all'uopo acquisite dall'azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud: ciò proviene sempre da parte della Giunta regionale campana. La medesima ASL Napoli 3 Sud ha colto l'occasione per assicurare che non risulta alcuna programmazione della chiusura del consultorio centro di neuropsichiatria infantile di Torre Annunziata, distretto sanitario n. 56. Lo stesso è regolarmente funzionante e non ha sospeso alcuna attività, data la rilevanza che rivestono le prestazioni sociosanitarie erogate nella struttura, che sono anzi state implementate. Sempre la Regione Campania ci dice dunque che le prestazioni sociosanitarie erogate nella struttura sono state implementate. L'ASL della Campania precisa che non sussistono dimensionamenti degli spazi occupati dalla neuropsichiatria infantile in quanto, a seguito del trasferimento del centro vaccinale consultoriale in una struttura maggiormente accessibile alla popolazione, sono state rese libere due stanze, una assegnata appunto alla neuropsichiatria infantile e l'altra impiegata per altre attività del consultorio e destinata ai corsi di preparazione al parto. Il personale del consultorio sopperisce alle carenze della neuropsichiatria infantile senza alcun depotenziamento delle varie attività sociosanitarie erogate. Così ci dice sempre la Giunta regionale della Campania, che ci riporta queste notizie, che non potremmo sapere diversamente, se non

dice che non sono vere, rinnovo il mio intendimento di essere al suo fianco, per la sanità pubblica e universalistica italiana. Più in generale, l'ASL Napoli Sud ha inteso sottolineare di aver ottemperato alle disposizioni regionali e di riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, di cui ai decreti del commissario *ad acta* del 22 settembre 2016, n. 99, avente ad oggetto il piano regionale di programmazione della rete per l'assistenza territoriale 2016-2018, e del 31 ottobre 2019, n. 83, piano regionale della rete di assistenza sanitaria territoriale 2019-2021. Detti decreti hanno delineato le modalità di erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza rivolte ai minori con problemi di salute mentale, disturbi del neurosviluppo e disagio psichico. La necessaria assistenza viene erogata tramite i nuclei di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NNPIA), che assolvono a molte delle attività in precedenza garantite dai servizi materno-infantili, che nel nuovo modello assistenziale della Regione Campania sono divenuti aree di coordinamento. Per garantire la continuità dei processi di cura, gli NNPIA vengono integrati nel dipartimento assistenziale per la salute mentale e hanno valenza sovradistrettuale. Napoli Sud in base al bacino di utenza sono stati definiti sei nuclei. Il nucleo 5 comprende il distretto sanitario n. 56 in questione, oltre al distretto sanitario n. 58, n. 58, e attualmente comprende tre medici specialisti neuropsichiatrici, uno specializzando, due psicologi, un logopedista, un assistente sociale e un infermiere. L'ASL Napoli 3 Sud è fortemente impegnata in un'azione di potenziamento della propria offerta assistenziale ed è protesa verso uno sforzo costante di implementazione degli NNPIA. In particolare, la stessa ASL dichiara di aver assunto neuropsichiatri, psicologi e logopedisti e sta procedendo a reperire altre figure professionali necessarie per la corretta erogazione della specifica assistenza. La ASL sta provvedendo anche al reperimento degli spazi idonei alle esigenze dei minori, del tutto diverse da quelle degli adulti e necessitanti di ambienti completamente separati da quelli destinati alla popolazione adulta. la sua risposta, che mi dà l'opportunità di fare un discorso anche più ampio.

però che, nel contesto di cui stiamo dibattendo, quello cioè dei servizi territoriali - in questo caso servizi di neuropsichiatria e precedentemente servizi di pronto soccorso, addirittura all'interno di un DEA di primo livello

Tale sistema non ha più una cabina di regia unica. E allora, oltre a fare una riflessione sul centro di neuropsichiatria o sul pronto sul pronto soccorso DEA di primo livello - in questo momento non funziona come tale, ma è fermo - dobbiamo anche capire se la cabina di regia funziona oppure no; se i livelli essenziali di assistenza e le garanzie costituzionalmente previste dall'articolo 32 esistono e sono davvero funzionali nei territori e nelle Regioni. infatti, andando avanti di questo passo, oggi non abbiamo queste tutele e domani, quando e se ci sarà un regionalismo differenziato in cui le singole Regioni vogliono altra autonomia,

la possibilità di avere presso il centro il contatto con il neuropsichiatra infantile. A pagarne le conseguenze sono stati i bambini disabili, i più piccoli, cioè i più fragili. In tutte le strutture ci sono differenti livelli di organizzazione e di *setting* ospedaliero - lo comprendiamo - ma il compito dello Stato

dal precedente problema dei DEA di primo livello, che non sono DEA, perché lei sa benissimo che per fare un DEA di primo livello serve un piano, un atto aziendale, che deve avere la firma del Presidente della Regione. tra l'altro, che questo atto aziendale di DEA di primo livello abbia la firma del presidente De Luca. Glielo dico, poi magari lo vedremo insieme, quando lei mi accompagnerà dal Presidente della Regione Campania e andremo a fare visita al DEA di primo livello, che non esiste, e al centro di neuropsichiatria infantile, che è stato demansionato e depotenziato.

di scendere a vedere quali sono i problemi del territorio e accompagnare dei processi di modifica, di trasformazione, utili a garantire la salute nei territori di cui sono rappresentante.

alle quali risponderanno il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso.

Quando, nella scorsa legislatura, con il Governo Draghi, il ministro Cingolani cominciò a parlare di nucleare, le forze che sostenevano quel Governo, che andavano dall'estrema sinistra alla Lega, ebbero diverse posizioni.

quando avete fatto la campagna elettorale e anche dalle sue prime interviste, sembrava che il tema fosse definitivamente sdoganato: il nucleare sembrava finalmente nell'agenda del Governo. E noi, oggettivamente, guardavamo con interesse a questa parte. chiedesse agli Stati europei di fare una strategia nucleare comune - anche perché, detto tra di noi, costerebbe anche di meno che non procedere come singoli Stati - e al tavolo del nucleare francese/europeo l'Italia non si è seduta. Quindi, noi siamo qui a chiederle come mai questo non è accaduto; se lo *slogan* del nucleare fosse solo uno *slogan* tal quale per la campagna elettorale o se effettivamente vi sia la volontà del Governo italiano di andare verso questa direzione. Anticipo una sua risposta. So che ci sono stati due *referendum* sul nucleare in Italia e ne conosco anche l'esito. Ma so anche che ENI, per esempio, sta procedendo nella ricerca sul nucleare pulito

In merito al quesito posto, vorrei sottolineare come l'atteggiamento positivo da parte dell'attuale Esecutivo verso il nucleare nasca da un approccio pragmatico, basato sul principio della neutralità tecnologica. Il nucleare di quarta generazione è una delle tecnologie da tenere in considerazione per affrancarsi dalle dipendenze dai combustibili fossili e, molto probabilmente, costituirà un vettore tecnologico di transizione propedeutico all'approccio finale, che è la fusione nucleare. Pertanto, l'Italia non può precludersi l'opportunità di proseguire nella ricerca in tale ambito, considerato inoltre che, negli ultimi decenni - come lei ha già avuto modo peraltro di rappresentare - abbiamo offerto alle Nazioni che hanno proseguito lo sviluppo del nucleare eccellenti professionisti e un *know how* che siamo pronti ad impiegare nella ricerca nei confini nazionali. Come già evidenziato durante l'illustrazione delle linee programmatiche, a livello internazionale si intende rafforzare la partecipazione dell'Italia nell'ambito del programma internazionale ITER e del programma europeo EUROfusion; così come sarà rafforzato il presidio scientifico nel campo degli impianti nucleari di quarta generazione e dei reattori modulari, gli *small modular reactor*. La mancata presenza di un rappresentante italiano all'iniziativa francese, informale, organizzata a margine del Consiglio energia e trasporti - peraltro ho anche parlato con il Ministro francese - rappresenta non un cambio di rotta dell'Esecutivo, ma semplicemente una forma permettetemi - di estremo rispetto della sovranità popolare del Parlamento italiano, il cui coinvolgimento è ritenuto essenziale da parte dell'Esecutivo prima dell'assunzione di impegni o prese di posizione a livello internazionale.

del Governo e del ministro Pichetto Fratin sul tema dello sviluppo della tecnologia del nucleare di quarta generazione siano generazione siano sicuramente condivisibili. Quindi, se il Governo ci dice che è interessato a seguire lo sviluppo della tecnologia e a partecipare ad azioni di impostazione europea

Il punto però, Ministro, rimane politico. Lei dice che quello era un incontro informale e io le rispondo che anche a un incontro informale il nostro Paese avrebbe dovuto partecipare per capire quale tipo di impostazione l'Europa vuole dare a questa soluzione, per non rimanere tagliato fuori. Vede, signor Ministro, l'isolamento del nostro Paese sul piano europeo con questo Governo sta diventando una cifra connotante: lo è su tanti temi e non vorrei che lo fosse anche sul tema dello sviluppo dell'energia e del nucleare, perché sarebbe un isolamento pesante, che rischieremmo di pagare in termini economici, produttivi e - mi faccia dire - anche ambientali. Quello Quello che voglio dirle, Ministro, è che sicuramente prendiamo atto del fatto che la vostra impostazione non è ostile al nucleare, ma la aspettiamo con i fatti e anche con il coinvolgimento del Parlamento, come lei giustamente ha detto; se il Ministro e il Governo vogliono coinvolgere il Parlamento e sfidarlo verso una soluzione utile al nostro Paese, lo faccia immediatamente. Non si perda altro tempo e non si perda il treno

nelle città metropolitane, da finanziarsi con i fondi della missione 2 del PNRR. A tale scopo, sono stati destinati 330 milioni con l'obiettivo di piantumare 6,6 milioni di alberi nel nostro Paese entro il 2024. Questo perché nei prossimi dieci anni è previsto che il 70 per cento della popolazione si trasferisca a vivere nelle nostre città, comportando inevitabilmente un vertiginoso aumento del consumo delle risorse naturali, che poi si trasforma in rifiuti, inquinamento e consumo massiccio del suolo, ancora di più rispetto a quanto già non avvenga nel nostro Paese. Quindi, l'aumento del verde urbano risulta necessario per tentare di mitigare queste conseguenze. Infatti, questi interventi sono finalizzati a preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici, ma anche a ridurre l'inquinamento atmosferico, grande piaga soprattutto al Nord, che ci pone in una situazione di infrazione europea già da molto tempo, con molteplici di uscire da questa situazione, che però non sanno sortendo i benefici auspicati. Gli interventi sono volti anche a recuperare paesaggi e a connessioni ecologiche (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) per valorizzare il sistema delle aree protette e frenare il consumo di suolo, come dicevamo anche prima. Le aree idonee per questi interventi devono avere caratteristiche ben definite, ma mi risulta - dalle segnalazioni che arrivano da alcune Città metropolitane - che ci siano talune difficoltà a identificare le aree adatte.

se abbiate pensato di adottare misure compensative per questi agricoltori, in modo da non generare squilibri occupazionali nelle sedi dove si vogliano piantumare gli alberi.

in merito alla questione posta dalla senatrice interrogante, riguardante l'investimento del PNRR denominato «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», si evidenzia che è stato emanato un primo avviso - pubblicato da parte del Ministero lo scorso 31 marzo 2022 - in cui, attese le specificità delle 14 Città metropolitane destinatarie della misura in termini di superficie-abitanti, complessità sociale ed economica, si è preferito lasciare margine di flessibilità in base alle diverse esigenze di ciascuna, individuando una superficie minima della proposta progettuale

Lo scorso 23 dicembre 2022 è stato raggiunto il *target* per il 2022, avendo ampiamente superato l'obiettivo di piantare almeno 1,65 milioni per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane, attraverso i 35 progetti ammessi a finanziamento. Il *target* successivo da raggiungere entro la fine del 2024 prevede la piantumazione di almeno 6,6 milioni di alberi. Al riguardo, è in corso di predisposizione il nuovo avviso per le annualità 2023 e 2024, in relazione al quale, in un'ottica di collaborazione istituzionale, è previsto un incontro con le Città metropolitane al fine di tener conto delle esperienze maturate nell'attuazione di questo primo avviso. Inoltre, è già stato previsto di apportare una serie di misure correttive finalizzate ad agevolare il reperimento delle aree stesse, come, ad esempio, la riduzione della superficie minima complessiva di progetto e la superficie minima della singola area di intervento. Infine, per quanto attiene alle eventuali misure compensative per gli agricoltori locatari dei terreni destinati alla piantumazione pubblica, è necessario evidenziare che tale tipologia di spesa non è ammissibile a valere sui fondi del PNRR. A questo riguardo sarà utile il confronto con i soggetti interessati, al fine di valutare eventuali soluzioni qualora le criticità evidenziate comportassero un rallentamento dei progetti di riforestazione urbana.

*(M5S)*. Signor Ministro, devo dirmi parzialmente soddisfatta della sua proposta. Mi pare di capire dalle sue parole che, comunque, qualche criticità è stata evidenziata anche al suo Ministero. Sono felice di apprendere che state cercando di porvi rimedio e mi auguro che riusciate in breve tempo ad arrivare a una soluzione in modo da poter effettivamente mettere a terra tutte quelle piante che ci servono tantissimo e che serviranno non solo per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche per creare quel microclima che faccia sì che aumentino anche le precipitazioni buone, ossia quelle che possono aiutarci a intervenire anche per quanto attiene alla crisi idrica senza avere quei fenomeni di bombe d'acqua a cui troppo spesso stiamo assistendo nel nostro Paese.

*(PD-IDP)*. Signor Ministro, desideriamo tornare sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, già affrontato recentemente in quest'Aula, proprio perché il recente annuncio della proposta di decreto, che disciplina gli incentivi all'autoconsumo, era atteso da tempo ma in forma molto più forte e con tempi certi. Ad oggi, non solo non si è sbloccato l'avvio delle CER, ma anzi ci è sembrato che siano stati ridimensionati il valore e la portata di questo strumento. Ricordo a noi tutti in quest'Aula le grandi potenzialità che hanno le comunità energetiche, poiché rappresentano una perfetta applicazione dei principi di sviluppo sostenibile. Esse infatti riescono a coniugare diverse aspetti: la responsabilità economica, poiché generano ricchezza sul lungo periodo sia per i partecipanti alla comunità energetica in termini di risparmio e ricavo, sia per le comunità locali e nazionale in termini di valore aggiunto; la responsabilità ambientale, considerato che svolgono un ruolo chiave nella transizione energetica; la responsabilità sociale, in quanto combattono la povertà energetica e promuovono lo sviluppo delle comunità locali anche nelle aree interne o economicamente più in difficoltà; e infine la responsabilità istituzionale, poiché promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali allo sviluppo e alla gestione del progetto. Quest'ultimo aspetto, troppo spesso ignorato, è essenziale, poiché non esiste sviluppo sostenibile senza una partecipazione attiva che trovi spazi e legittimità in un assetto istituzionale riconosciuto. Ma di fronte ai ritardi a cui abbiamo assistito, alle lungaggini burocratiche, alla mancanza fino ad oggi degli incentivi da parte del Ministero, al ritardo di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo, ci chiediamo: il Governo crede davvero nelle comunità energetiche e nello sviluppo sostenibile? Per comprenderlo, le poniamo quindi tre questioni precise, sperando di avere da lei risposte altrettanto precise. La prima: qual è l'avanzamento delle interlocuzioni con la Commissione europea e quando, di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che entrerà in vigore il decreto che disciplina gli incentivi? La seconda: intende il signor Ministro attivarsi con nel rispetto delle reciproche prerogative istituzionali ma con tutto il peso del suo ruolo, affinché ARERA adotti finalmente le misure con le quali i clienti domestici possano richiedere lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa? Infine, non ritiene opportuno e urgente adottare un piano nazionale per il risparmio energetico per interventi finalizzati ad aumentare drasticamente la quota di rinnovabili prodotta in Italia; un piano da affiancare alle misure già previste al fine di garantire un più rapido raggiungimento da parte del nostro Paese degli obiettivi di sviluppo e diffusione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico e, conseguentemente,

come già annunciato nella seduta di *question time* al Senato della scorsa settimana, la proposta di decreto sulle comunità energetiche e sulle configurazioni di autoconsumo, che contempla sia lo schema di incentivazione previsto dall'articolo 8 del decreto n.199 del 2021, sia l'attuazione della misura prevista nel PNRR, è pronto. La sua entrata in vigore è subordinata unicamente all'approvazione della Commissione europea, con cui sono state certamente avviate le interlocuzioni, ma la determinazione dei tempi è da parte della Commissione. Questo provvedimento pone al centro delle scelte energetiche del Paese le comunità e e al contempo ha l'effetto benefico di rivalorizzare i territori e aumentare la consapevolezza dei membri sull'autoconsumo di energia da fonti *green.* Secondo gli analisti - spero sia così - si dovrebbero superare le 15.000 comunità. Con la misura, si intende incentivare la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili per un contingente di potenza complessiva fino a 7.000 megawatt entro il 2027, obiettivo che penso raggiungeremo prima. Il Ministero avvierà inoltre apposite iniziative e campagne informative al fine di garantire ai cittadini un'adeguata informazione sui benefici derivanti dall'adesione a una delle configurazioni e sulle modalità con le quali massimizzare l'autoconsumo, al quale è legato il riconoscimento dell'incentivo in tariffa, e cumulare anche il contributo in conto capitale previsto dal PNRR nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ricordando che lo stanziamento è di 2 miliardi e 200 milioni. Per quanto concerne un piano nazionale per il risparmio energetico, auspicato dai senatori interroganti, si deve rilevare che il panorama nazionale già contempla diverse azioni volte al contenimento dei consumi energetici, che vanno dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di prossimo aggiornamento, al Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, sino all'insieme delle misure e dei benefici fiscali per gli interventi di efficienza energetica e recupero del patrimonio edilizio esistente. Infine, le misure di semplificazione per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili previste dal decreto-legge PNRR sono ora al Senato e contribuiranno al ribaltamento dell'attuale rapporto di utilizzo delle fonti di energia,

nell'emanazione dei decreti di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, che oggi non le hanno consentito ancora di poterci fornire una data certa, perché solo recentemente sono stati comunicati alla Commissione europea. La decisione di non portare avanti un piano nazionale per il risparmio energetico, ma di continuare ad avere più misure, come quelle che lei ci ha descritto, crediamo che non sia la scelta che serve in questo momento al Paese. Non è comprensibile, da parte nostra, la scelta di non mettere al centro l'idea di un piano per le energie rinnovabili e l'autoproduzione come cardine di una nuova politica energetica.

che ha questa sfida. Crediamo, ribadiamo e speriamo con questa nostra interlocuzione di aver dato un segnale perché si rimetta al centro un piano rivolto alle energie rinnovabili e all'idea di comunità energetiche come maggior risposta a quella che in questo momento è una grande sofferenza del Paese, cioè la povertà energetica. L'idea della comunità energetica non si fonda infatti sull'idea degli incentivi, ma, partendo dagli incentivi, permette di costruire un vero e proprio piano industriale che poi funzioni con le proprie gambe e possa dare una risposta al Paese. Crediamo che sia un vero e proprio intervento di politica industriale ed energetica quello che serve all'Italia, che non incentivi le fonti fossili, ma acceleri la transizione. Questo è quello di cui - secondo noi - ha bisogno in questo momento il nostro Paese.

Signor Presidente, colleghi, gentile Ministro, oggi in Aula sottopongo all'attenzione del Governo il tema dei dottorati. L'Italia è uno dei Paesi OCSE con il più basso tasso di studenti di dottorato. L'ultimo rapporto Education at a Glance 2022 registrava,

solo lo 0,5 per cento della popolazione in età lavorativa in Italia ha un dottorato di ricerca. In Europa la stessa percentuale, in media, è dell'1,2 Il numero di dottorandi è significativo per un Paese che vuole sfruttare al meglio la propria capacità di creare innovazione e quindi di guardare al futuro. Sappiamo tutti quanto sia importante la sfida del PNRR. Per sfruttarla al meglio è però necessario affiancarle un patto delle competenze. Cito un dato: nel 2022, il 43 per cento delle assunzioni programmate dalle aziende italiane non è andato a buon fine per mancanza di profili adatti. Lo *skill mismatch* tra domanda e offerta di lavoro è una realtà che, per il Governo e la maggioranza, rappresenta una priorità da affrontare. Su questo aspetto, il PNRR non a caso prevede un impegno rilevante per colmare lo *skill gap*, cruciale per sostenere un ecosistema dell'innovazione. I bandi del PNRR per borse di dottorato, per un totale di 7.500 posti, rappresentano un primo e significativo passo in avanti. Bisogna fare di più: il 2023 rappresenta un anno chiave per voltare pagina. Servono un significativo incremento in termini di risorse finanziarie, nel sostenere nuove borse di dottorato, e incentivi specifici per rendere più attrattive le prospettive di lavoro dei futuri dottori

sono nei principali *ranking* internazionali. Bisogna avvicinare il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Le risorse del PNRR ci sono e vanno bene. Il PNRR è una scintilla, ora dobbiamo alimentarla. Come? Sfruttando bene le risorse e investendo sui dottorati innovativi, guardando ad un disegno che abbia una prospettiva e una visione di almeno venti Per questo motivo pongo oggi all'attenzione del Governo la seguente importante e fondamentale questione. Al ministro Bernini, che ringrazio per essere qui con noi, oggi pomeriggio, chiediamo come l'Esecutivo intenda intervenire per agevolare il raggiungimento di *target* impegnativi e al tempo stesso strategici per il Paese, rendendo maggiormente attrattivi i percorsi di dottorato, sia in generale, sia in modo particolare quelli innovativi, che guardano al mondo produttivo.

Sono io che ringrazio il presidente De Poli per aver posto l'attenzione sul tema dei dottorati di ricerca e anzi sul tema dei dottorati, della ricerca e dell'impresa, a cui come Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale attribuiamo un ruolo centrale, anzi strategico per la vita del Paese.

In questa prospettiva, il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che lei evocava, potrà essere determinante per la crescita esponenziale dei numeri da lei indicati. Grazie anche alle risorse assicurate dal Piano sarà possibile agire su due livelli distinti, con il risultato di valorizzare i percorsi dei dottorati e i loro sbocchi occupazionali: questa è in assoluto la cosa più importante. Il nostro primo obiettivo è garantire un adeguato supporto finanziario per un numero sempre crescente di borse di studio. Su questa linea di intervento le do una notizia, presidente De Poli: ho firmato proprio ieri due decreti ministeriali che assicurano 18.770 borse di dottorato, con un finanziamento di oltre 726 milioni di euro. Le borse di dottorato di ricerca saranno bandite per il prossimo anno accademico 2023-2024, quindi subito. Al tempo stesso stiamo lavorando per accrescere l'attrattività di questi percorsi, proprio in relazione alle prospettive occupazionali, mettendoli in stretta relazione con il mondo produttivo e, quindi, rendendoli attrattivi per le imprese. In questa direzione, con il decreto-legge n. 13 del 2023, il cosiddetto decreto PNRR, sono stati introdotti benefici contributivi a favore delle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo e che puntano ad un innalzamento delle qualifiche del personale. Potranno infatti giovarsi del taglio del cuneo fiscale per l'assunzione di dottori di ricerca per un investimento complessivo pari a 150 milioni di euro, messi a disposizione dal PNRR, per agevolare un totale di 20.000 assunzioni. Sono numeri reali, presidente De Poli. L'obiettivo è creare un circolo virtuoso che abbia, a monte, esperienze di cofinanziamento tra pubblico e privato e, a valle, incentivi all'assunzione di personale qualificato. È così che puntiamo a far emergere il legame imprescindibile tra ricerca e impresa, investendo nel capitale umano e creando un sistema nazionale della ricerca basato sulla capacità di fare rete tra università, enti di ricerca e imprese. Sarà nostro compito, con il vostro aiuto, fare in modo che non vi siano più occasioni mancate e che l'Italia si allinei agli *standard* degli altri Paesi europei. Signor Ministro, mi ritengo piacevolmente soddisfatto dalla sua risposta e non in quanto senatore di quest'Aula della Repubblica italiana, ma soprattutto per i giovani,

anche lei. Un altro aspetto altrettanto positivo è il taglio del cuneo fiscale per chi assume e fa un percorso con i dottori di ricerca: anche qui 20.000 assunzioni con il cofinanziamento.

Ministro, come sappiamo bene, con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 1999, il sistema universitario italiano ha adottato il numero chiuso programmato per disciplinare l'iscrizione ad alcune facoltà. Numerose università hanno deliberato l'introduzione del numero chiuso per molti corsi. Sappiamo altresì che attorno ai *test* di accesso si è sviluppato negli anni un fiorente mercato di assistenza legale, a causa di vari ricorsi avviati al TAR nelle varie Regioni d'Italia, nonché costosi corsi privati di preparazione, con la conseguenza di un onere per le famiglie italiane, le quali si vedono discriminate ulteriormente di fronte al fondamentale diritto all'istruzione pubblica; un diritto, peraltro, sancito e riconosciuto dalla Costituzione italiana. Crediamo, peraltro, che, di fronte alla crescente disoccupazione giovanile, sia sempre più necessario intervenire in istruzione e in formazione, garantendo uguali possibilità di accesso allo studio così come alla ricerca di un posto di lavoro. Sappiamo anche che molti giovani si recano all'estero, per esempio, per i corsi di medicina e di odontoiatria, soltanto per conseguire la laurea, aggirando in questo modo la normativa italiana che prevede i numeri programmati, e che i corsi di laurea in scienze della formazione sono insufficienti a laureare un numero adeguato di maestri abilitati e corrispondenti al fabbisogno reale

degli aspiranti iscritti o richiedono conoscenze assai specifiche. La prassi, peraltro, ha prodotto molteplici effetti: un numero rilevante di studenti ripiega verso facoltà nelle quali non è previsto il numero chiuso; altri decidono per l'iscrizione ad atenei stranieri e altri ancora si vedono costretti a rinunciare agli studi. Noi pensiamo che la necessità di premiare il merito debba essere un elemento di selezione durante il percorso di studi, ma non nell'accesso ad esso. Le chiedo pertanto se intende promuovere la modifica di queste disposizioni, al fine di evitare di assistere alla continua emigrazione di risorse umane qualificate che scelgono di lavorare e produrre al di fuori del nostro Paese; intende attivarsi al fine di abolire il test di medicina. Naturalmente, in questo caso, le chiedo quali azioni in alternativa intende promuovere al fine di garantire il libero accesso alla formazione universitaria e al diritto allo studio, per esempio incrementando i fondi per aumentare i docenti di riferimento dei corsi di laurea necessari a non abbassare il livello di qualità degli studi secondo i parametri vigenti. PRESIDENTE.

De Cristofaro non solo per aver affrontato il tema dell'accesso programmato ai corsi di laurea, ma anche per averlo fatto con un approccio ampio e propositivo, coinvolgendo anche profili non sempre oggetto di opportuno approfondimento. In particolare, ho apprezzato il riferimento alla qualità dei percorsi formativi; troppo spesso, invece, ci si concentra solo sul livello quantitativo dell'accesso ai corsi di studio. L'accesso programmato ai corsi di studio non è tanto e solo pensato per limitare il numero delle immatricolazioni, né solo per ridurre il numero dei laureati perché sproporzionato rispetto alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro. Si tratta in parte di mantenere uno *standard* qualitativo adeguato e costante nei percorsi di formazione, specie per quei profili professionali per i quali si richiede un'integrazione tra didattica frontale ed esperienze di tirocinio. la programmazione degli accessi va analizzata da due punti di vista, come l'interrogante ha giustamente evidenziato: da un lato, alla luce delle esigenze del fabbisogno di personale; dall'altro, in relazione alla capacità didattica e formativa che gli atenei sono in grado di assicurare, mediante l'integrazione tra attività didattiche ed esperienza pratico-applicativa anche valorizzando il tessuto territoriale di prossimità. La previsione di un numero predeterminato di posti disponibili è in alcuni ambiti opportuna, così da mantenere alta la qualità della formazione e ridurre il più possibile il solco tra domanda e offerta di professionalità, avvicinando il profilo in uscita dal percorso formativo a quello richiesto per l'immissione al mondo lavorativo professionale. Vorrei dire con molta chiarezza che il livello di programmazione non può essere commisurato alle capacità formative del sistema - questo sarebbe un sacrificio per gli studenti - sulle quali anzi bisogna agire per finanziarle e rafforzarle. La sfida che ci siamo posti è individuare un livello sostenibile degli accessibili che assicuri maggiori ingressi legati al fabbisogno progressivo, senza per questo trascurare la qualità della formazione. Non ci possiamo permettere di fare neanche questo. Questo è il criterio che sta guidando i lavori in corso sull'apertura sostenibile degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e che dovrà - secondo noi - costituire un modello per una rilevante manutenzione della legge n. 264 del 1999 sull'accesso programmato.

Non sono ancora soddisfatto del tutto, perché credo che servirebbe ancora maggiore coraggio per portare avanti una questione che penso essere oggi di pienissima attualità, per l'appunto il superamento pieno del numero chiuso. Esiste naturalmente il tema della qualità lei stessa ha riconosciuto che io ne ho voluto parlare nell'interrogazione. Esiste anche un tema che riguarda - l'abbiamo visto anche durante la pandemia - una carenza strutturale di medici e di odontoiatri in questo Paese. Pensiamo Pensiamo che da questo punto di vista sia obiettivamente utile per tutti affrontare la questione il più rapidamente possibile. So che esiste una commissione e spero che possa svolgere possa svolgere un lavoro. So anche che il meccanismo è cambiato rispetto al passato: adesso - come sappiamo - i *test* si fanno o comunque si faranno più volte nel corso del tempo, già a partire dal penultimo anno delle scuole superiori. Non sono convintissimo, in verità, che questa sia la soluzione e, anzi, temo che una tale metodologia possa addirittura aumentare il livello di competitività e finanche lo *stress* emotivo di chi poi il *test* va a fare. In ogni caso, voglio chiudere il mio intervento con un tema che penso debba essere quanto più trasversale possibile e spero quanto più condiviso possibile. Credo che, per superare il numero chiuso o comunque le difficoltà che ci sono state in questi anni, o anche per esempio per superare il cosiddetto imbuto formativo per la specialistica, che è l'altro grande problema che lei conosce perfettamente, servano investimenti strutturali di lungo periodo. Quindi si torna sempre al principale problema: il nostro Paese in questi anni ha investito poco sulla scuola, sull'università e sulla ricerca. Se si investisse invece molto più di quello che è stato fatto, credo che potremmo trovare delle soluzioni, anche e soprattutto per risolvere le questioni di cui abbiamo parlato oggi. La ringrazio in ogni caso molto per la risposta.

della ricerca* - Premesso che: le prove di ammissione per l'accesso ad alcuni corsi universitari sono state istituite allo scopo di consentire agli atenei di organizzare i corsi di laurea secondo parametri più prossimi a quelli in uso in Europa e nel resto del mondo. Per quanto riguarda però soprattutto la facoltà di medicina, sono troppi gli studenti penalizzati che non riescono a soddisfare le proprie scelte formative. La politica e la programmazione sanitaria in termini di personale faticano a reperire nuove risorse per garantire la formazione a giovani medici che sostituiscano quelli in uscita per quiescenza. Secondo una stima di Anaao Assomed, uno dei principali sindacati di medici ospedalieri, entro il 2024 mancheranno almeno 40.000 medici a causa della programmazione sbagliata nel tempo. Negli anni scorsi, numerosi sono stati i ricorsi presentati da studenti che contestavano non solo l'esito della loro prova di ammissione, ma anche la sua adeguatezza in termini di effettiva conformità al tipo di facoltà alla quale intendevano iscriversi. Infatti, molti dei *test* che venivano somministrati non erano parametrati sulle materie attinenti alle facoltà scelte dai candidati, ma riguardavano argomenti del tutto estranei. Da un'analisi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca era emersa la necessità di rivedere i criteri di analisi utilizzati allo scopo di garantire i necessari livelli qualitativi degli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari. Ecco perché nel 2023 il *test* è cambiato completamente. Si tratta di un esame TOLC, ovvero di un *test* di orientamento per l'ingresso all'università; il *test* si può ripetere più volte l'anno a partire dal quarto anno delle superiori e il Ministero stabilisce una data in cui tutti i candidati devono registrare il migliore dei risultati ottenuti, così da definire la graduatoria nazionale e, in base ai posti disponibili degli atenei, assegnare gli spazi, tenendo conto delle preferenze indicate dai candidati. Da una attenta analisi della normativa europea in materia non vi è traccia di una imposizione del numero chiuso. L'Unione europea chiede solo di armonizzare i sistemi formativi e gli *standard* di qualità, affinché i professionisti possano muoversi liberamente nello spazio europeo del lavoro vedendo riconosciuti i propri titoli. In Italia, il numero chiuso è regolato dalla legge n. 264 del 1999, approvata per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998, con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi al numero programmato, per disciplinare la materia. Il sistema dei *test* d'ingresso alle facoltà universitarie, oltre ad incidere pesantemente sul diritto allo studio costituzionalmente garantito, per quanto attiene particolarmente alla facoltà di medicina e chirurgia sta letteralmente decimando la classe medica del futuro, costringendo il nostro Paese a importare importare medici da Paesi stranieri, come già avviene da anni nel settore infermieristico. Si chiede, quindi, a lei, signor Ministro, stante la situazione emergenziale ampiamente descritta in premessa, quali misure siano allo studio per arrivare a soluzioni che consentano di aumentare il numero dei posti disponibili alla facoltà di medicina, preservando, al contempo, la qualità dell'insegnamento, anche in considerazione della necessità,

ringrazio il presidente Marti e tutto il Gruppo parlamentare della Lega per questa occasione di confronto su un tema tanto sentito, che considero assolutamente caratterizzante il lavoro del Ministero dell'università e della ricerca e l'attività del Governo nel suo complesso. Il lavoro in corso sugli accessi alla laurea in medicina e chirurgia è in atto da tempo e anche recentemente vi sono stati interventi di modifica, che lei, presidente Marti, correttamente ricordava. A partire dall'anno accademico 2022-2023, quindi ora, si è passati a nuove modalità di esame (TOLC), ripetibili più volte e accessibili già agli studenti iscritti al penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Si è trattato di una modifica interessante, che tra l'altro ha già avuto buoni risultati nei corsi ai quali è stata applicata, ad esempio ingegneria. Anche qui, però, vorrei essere molto chiara e dire che, da sola, essa non può risultare soddisfacente. Il tema resta aprire i numeri di accesso a medicina, adeguandoli al fabbisogno reale di medici e di specialisti nel tempo; il tutto anche in considerazione dei prossimi pensionamenti di medici attualmente in attività e del progressivo - per fortuna - invecchiamento della popolazione. Il 12 gennaio scorso siamo partiti con un lavoro focalizzato sulla apertura programmata degli accessi; lavoro che coinvolge non soltanto noi e il Ministero della salute, ma anche le Regioni e le università, nonché, attraverso contributi importantissimi di consultazione, le categorie professionali. Il lavoro in corso punta a definire il fabbisogno dei medici e ad adeguare la capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario, al fine di rivedere i meccanismi di programmazione degli accessi, nel senso dell'apertura ovviamente.

preservando il livello qualitativo della formazione, che richiede la valorizzazione dello svolgimento di internato nei reparti, e promuovendo il rafforzamento delle opportunità di tirocinio, anche in convenzione con le aziende ospedaliere; per aprire l'università ai territori e modellare il fabbisogno del personale sanitario alle esigenze delle realtà territoriali. Miriamo, dunque, ad un accesso sostenibile, ad una apertura sostenibile delle professioni sanitarie,

Tutto questo da subito, a partire dalla chiusura del tavolo, che avverrà intorno al mese in confronto con le Regioni e la CRUI, che è la *Conferenza* dei rettori delle università italiane, individuando poi, di conseguenza, il numero degli accessi necessari per colmare esattamente il *gap* - da lei ricordato correttamente - ad oggi esistente. Signor Presidente, signor Ministro, siamo soddisfatti della sua risposta, dalla quale si evince che finalmente, dopo anni di critiche al sistema e ricorsi, si sta procedendo ad un cambio di regime degli accessi alla facoltà di medicina. Da anni la Lega e Matteo Salvini auspicano una revisione dell'accesso alle professioni mediche per assicurare a tutti gli studenti il diritto allo studio e seguire le proprie aspirazioni professionali. Come ha già sottolineato, auspichiamo che quella che è emersa dal confronto con le Regioni, che per ora riteniamo una prima stima prudenziale nelle percentuali di aumento degli accessi alla facoltà di medicina, potrà essere poi riconsiderata, sapendo tutti che i primi successi si avranno fra sei-otto anni

sappiamo che lei è alla guida della più grande impresa italiana per numero di dipendenti, la pubblica amministrazione, che ne conta circa 3,2 milioni. Ovviamente parliamo di tutti i dipendenti pubblici, quelli impegnati in ruoli più specializzati, come medici, insegnanti e vigili del fuoco, che rendono servizi che si vedono e possiamo anche apprezzare, ma parliamo anche di tanto personale amministrativo, la cui presenza è legata alle troppe incombenze previste da quel largo tessuto di leggi e decreti che guidano le tante procedure per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Alcuni fatti di cronaca evidenziano che, nonostante gli sforzi finora sostenuti, la relazione tra cittadini, imprese pubbliche e amministrazioni appare ancora difficile. La pandemia, con il distanziamento sociale e i limiti agli orari di apertura al pubblico degli uffici, accentuato alcune problematiche nell'accesso ai servizi. La maggiore criticità deriva dalla difficoltà da parte degli utenti nella segnalazione di eventuali inadempienze delle amministrazioni pubbliche. Per capire come far funzionare meglio la macchina pubblica, lei ha cominciato a girare i territori con in testa l'idea di far semplice l'Italia: questo prevede una sorta di controllo di gestione, con lo scopo di dare maggiore trasparenza all'intera azione amministrativa, ma è necessario anche riuscire a semplificare tutte quelle procedure, spesso eccessive, che potrebbero essere sostituite da procedure elettroniche, o addirittura eliminate, laddove superflue o ripetitive. quindi un grande lavoro di individuazione delle esigenze dei cittadini e, al contempo, l'ascolto della necessità dei lavoratori della pubblica amministrazione, che giustamente hanno rivendicazioni da portare avanti. Questo premesso, le chiediamo, signor Ministro, se non intenda sviluppare le opportune iniziative volte a prevedere strumenti idonei a facilitare la relazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese e per implementare servizi sempre più efficienti.

che mi viene data di affrontare un tema che considero cruciale e riguarda nello specifico il rapporto tra gli utenti, cittadini e imprese, e le pubbliche amministrazioni. A questo proposito, voglio raccontarvi che da dicembre 2022 è *online*, in via sperimentale, il portale «LaTuaPA», che consente a ogni cittadino di segnalare presunte irregolarità e inadempienze delle amministrazioni, promuovendo, attraverso l'intervento dell'Ispettorato della funzione pubblica, la risoluzione delle criticità. Autenticandosi con SPID, con il Sistema pubblico di identità digitale, attraverso pochi e semplici passaggi, gli utenti possono inviare segnalazioni su ciò che non va nella pubblica amministrazione e seguire lo stato di avanzamento del procedimento e il suo esito. In sintesi, questo portale intende intanto rispondere all'esigenza di migliorare il rapporto con i cittadini, le imprese e le altre amministrazioni, garantendo efficienza e trasparenza della procedura; semplificare e velocizzare il lavoro dell'Ispettorato, attraverso la completa digitalizzazione delle istanze; infine, supportare i processi decisionali attraverso la produzione di informazioni dettagliate in ordine alle criticità riferite all'azione della pubblica amministrazione emerse nel corso dell'attività ispettiva. In questi primi due mesi di sperimentazione del portale, già un terzo delle segnalazioni all'ispettorato per la funzione pubblica è pervenuto proprio attraverso questo nuovo canale di comunicazione digitale e, nello stesso periodo, sono stati poco più della metà i procedimenti conclusi tra quelli complessivamente trattati sulle presunte irregolarità o inadempienze delle pubbliche amministrazioni. Andando ancora più nel dettaglio, in due mesi sono state 792 le segnalazioni trattate, di cui 260 relative a verifiche già in corso prima dell'avvio della piattaforma e altre 530 sono state acquisite successivamente. Rispetto al totale delle segnalazioni trattate, nel 50 per cento dei casi il procedimento è stato concluso; quanto ai procedimenti in fase di istruttoria, nel 17 per cento dei casi è già stata avviata una verifica presso la pubblica amministrazione segnalata, e in generale va rilevato che la maggior parte del complesso delle segnalazioni, pari quasi al 90 per cento, riguarda presunte inadempienze della pubblica amministrazione cui è connessa la lesione di un interesse particolare del cittadino, mentre per il restante 12 per cento si fa riferimento a presunte irregolarità dell'azione amministrativa cui è connessa la lesione di interesse di portata generale. L'implementazione del portale sta rafforzando l'attività di ascolto dei cittadini con le amministrazioni pubbliche, lasciando emergere criticità più ricorrenti di servizi riscontrati dei cittadini. In questo modo, promuovendo un modello di amministrazione sempre più aperta, trasparente e vicina agli utenti, saremo capaci non solo di verificare e misurare il grado di efficacia del lavoro delle amministrazioni, ma soprattutto di correggere eventuali disfunzioni emerse nell'attività di controllo. In conclusione,

ci sentiamo veramente fieri di questa sua risposta e siamo anche convinti che, venendo lei dal mondo del lavoro, è l'uomo giusto al posto giusto, che riesce a motivare i lavoratori della pubblica amministrazione e non solo loro, anche i clienti, che sono i cittadini e le aziende. Le auguro di continuare così e la ringrazio. *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, una domanda che ci viene rivolta con tanta frequenza - lei sicuramente non è da meno nell'ambito del lavoro: tutti ci chiedono notizie di questo o quel concorso piuttosto che di questa o di quella graduatoria, nel mondo delle Forze dell'ordine, della giustizia o della sanità; e naturalmente, non poteva mancare il mondo della pubblica amministrazione. Quindi, quale persona meglio di lei ci può rispondere nel merito? merito? Chiediamo quindi direttamente a lei, considerato che da un *forum* della pubblica amministrazione 2022, durante il quale è stata presentata la ricerca sul lavoro pubblico, è emerso che entro il 2028 - quindi, da qui ai prossimi cinque anni - serviranno oltre 800.000 assunzioni. In Italia oggi ci sono meno lavoratori pubblici rispetto agli altri Paesi europei, una pubblica amministrazione anziana, con un'età media di cinquant'anni, purtroppo scarsamente aggiornata; le medie parlano di poco più di un giorno di formazione per ogni dipendente all'anno. Sono in difficoltà nell'offrire servizi adeguati a imprese e cittadini. Da un sondaggio emerge che il 70 per cento degli italiani, purtroppo, li considera inadeguati, mentre gli europei sono insoddisfatti quasi al 51 Il «Sole 24 Ore» riporta il *report* di ForumPA e dice che al 1° gennaio 2021 la nostra pubblica amministrazione contava 3,2 milioni di dipendenti, 31.000 in meno rispetto all'anno precedente: abbiamo toccato il minimo storico negli ultimi vent'anni. Dopo un timido segnale di crescita del personale nel 2020, il blocco dei concorsi causato dall'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non hanno permesso al *turnover* di ritrovare l'equilibrio sperato. Al 1° gennaio 2022, infatti, erano poco più di 3 milioni i pensionati dal lavoro pubblico. Tale esodo è destinato, purtroppo, ad aumentare, come descritto nello stesso rapporto del ForumPA. Nel prossimo triennio almeno 300.000 persone del pubblico impiego andranno in pensione, ma probabilmente saranno molte di più, se consideriamo oltre 500.000 dipendenti che hanno oltre sessantadue anni e più di 180.000 di loro hanno raggiunto i trentott'anni di anzianità di servizio, per cui parliamo complessivamente di circa un milione di pensionati. Nonostante i dati impietosi, la pubblica amministrazione è chiamata ad essere il motore della ripresa disegnata con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo stesso Ministro interrogato, con riferimento all'evoluzione degli organici della pubblica amministrazione, ha più volte annunciato che nel 2023, sulla scia di quanto già iniziato nel 2022, quando sono stati immessi in ruolo circa 157.000 statali, il Governo garantirà una crescita del personale nella pubblica amministrazione, con oltre 156.000 nuove assunzioni, sottolineando come la pubblica amministrazione non abbia bisogno solo di numeri, ma di conoscenze e competenze da valorizzare al massimo. Un caso emblematico è quello del concorso unico lavoro Ripam, bandito nel 2019 e tenutosi nel 2021, a causa delle misure di contenimento dei contagi da mirava all'assunzione di 850 figure di funzionario da ripartire presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad oggi, della relativa graduatoria residuano circa 4.500 soggetti idonei a occupare posti da funzionario. Chiediamo di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per favorire il rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione; se intenda avvalersi del meccanismo dello scorrimento delle graduatorie dei soggetti risultati idonei, come ad esempio nel caso del concorso unico lavoro Ripam di cui in premessa, o permettendo che alla medesima graduatoria possano attingere altre amministrazioni interessate ad avvalersi di risorse già selezionate. PRESIDENTE. Il ministro per la pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, onorevoli senatori, mi ponete due quesiti che richiederebbero molto di più dei tre minuti che mi sono concessi per rispondere e quindi cercherò di fare di necessità virtù. La pandemia prima e il Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo ci hanno fatto capire quanto effettivamente sia strategico per il nostro Paese disporre di una pubblica amministrazione efficiente e rapida, digitalizzata, dotata di personale motivato e adeguatamente formato, capace di dare ai cittadini e alle imprese le risposte che chiedono in tempi rapidi e in modalità certe. Per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, dobbiamo innanzitutto puntare su un reclutamento di qualità per selezionare capitale umano qualificato e cercare di mettere le persone giuste al posto giusto. Gli anni antecedenti alla pandemia hanno visto, a causa delle politiche di contenimento della spesa pubblica - voglio ricordare che dal 2009 al 2019 c'è stato il blocco del *turnover* per cercare di rispettare il patto di stabilità di stabilità - un progressivo indebolimento delle pubbliche amministrazioni che si è riflesso negativamente in termini di investimenti in persone, di competenze e di innovazione organizzativa. Oggi abbiamo il dovere - lo dico innanzitutto a me stesso - e la possibilità di invertire questo *trend.* Basti pensare, come confermato dai dati forniti dagli onorevoli interroganti - l'ha ricordato appena lei nel suo quesito - che nel 2022 abbiamo inserito 157.000 persone e altrettante ne inseriremo nel 2023, quindi stiamo parlando di linfa vitale su cui le amministrazioni possono contare. Si tratta della possibilità di introdurre nel sistema pubblico personale giovane, qualificato e motivato, reclutato con procedure innovative. Abbiamo avviato a gennaio il portale InPA, gennaio il portale InPA, completamente digitale, per la gestione dei concorsi pubblici, e un nuovo regolamento, che approderà peraltro al parere delle Commissioni parlamentari dopo il passaggio che è tuttora in corso al Consiglio di Stato; e poi, attraverso la valutazione non più soltanto delle conoscenze, ma anche delle competenze trasversali, a breve pubblicheremo linee guida destinate alla selezione del personale non dirigenziale, mentre quelle per il personale dirigenziale le abbiamo già adottate lo scorso anno. Non basta reclutare, lo ricordava anche lei senatore, ma dobbiamo anche recuperare un *gap* formativo che si è accumulato in questi anni di *spending review.* Dobbiamo destinare le risorse necessarie a finanziare tutte le attività che concorrono alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla qualificazione del personale in servizio nella pubblica amministrazione. Voglio ricordare che stiamo attraversando anche una fase di trasformazione digitale che ci impone la necessità di avere un'attenzione alla formazione delle nostre persone. Lei ricordava esattamente che oggi i nostri dipendenti pubblici hanno un giorno di formazione all'anno, che personalmente considero assolutamente insufficiente. Con riguardo invece al secondo quesito, evidenzio che le pubbliche amministrazioni possono già assumere nuovo personale, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti. In particolare, le graduatorie vigenti dei concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, tra cui il concorso unico lavoro, sono rese disponibili alle amministrazioni che richiedono di attingervi per l'assunzione di nuovo personale. A conferma di ciò, proprio con riferimento al concorso da lei indicato, nello scorso mese di febbraio si è provveduto a fornire immediato riscontro alle amministrazioni richiedenti per l'attingimento di 794 nuove unità da assumere. In particolare, posizioni si è provveduto allo scorrimento della graduatoria del profilo di ispettore del lavoro, mentre per 247 si è dato corso allo scorrimento della graduatoria del profilo di funzionario di area amministrativa giuridico-contenziosa. PRESIDENTE. Ha facoltà Grazie, signor Ministro. Naturalmente, non ci poteva essere risposta migliore di questa per un'interrogante come me, in rappresentanza del partito. Ringraziamo il Governo per tutto il lavoro che sta facendo. Sappiamo anche che domani, a seguito di un altro concorso che si è svolto, lei ha dato la disponibilità a incontrare quanti vi hanno partecipato, i quali finalmente, dal luglio 2022, hanno visto la graduatoria forse qualche giorno addietro; anche loro sono fiduciosi del lavoro che si sta facendo. Naturalmente, il Governo sta lavorando nell'ambito nel mondo del lavoro; l'abbiamo dimostrato con l'approvazione del decreto milleproroghe, allorquando abbiamo approvato emendamenti che riguardano sia la sanità, con il reclutamento del personale sanitario e amministrativo che ha lavorato durante il periodo del Covid,